del ministro La Russa, che assume di aver voluto difendere l'onore dei militari italiani, ci sembrano superflue: l'onore dei militari italiani è fuori discussione e fortunatamente non è nella disponibilità del Ministro *pro tempore*.

quest'Aula sui fatti inerenti il respingimento avvenuto circa una settimana fa. Questa è la nostra richiesta. Sarà quella la sede per affrontare anche le dichiarazioni del ministro La Russa e le conseguenze che esse hanno determinato. *(Applausi

Ci auguriamo anzi che l'attenzione a questi temi ci consenta di esaminare ed approvare rapidamente il disegno di legge sulla sicurezza, che contiene norme di grande utilità ed importanza;

ha agito ed agisce sulla base delle norme del diritto internazionale e sulla base degli accordi che sono stati sottoscritti nel passato e rafforzati recentemente

contrario, nel rispetto delle promesse che abbiamo fatto in campagna elettorale e tenendo conto di quello che ci chiede la gente, noi vogliamo finirla per sempre con l'immigrazione clandestina in questo Paese

nelle tribune gli studenti dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «Ercole Rosa» di Sarnano (Macerata). A loro rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio e la conclusione dell'anno scolastico.

come è a tutti noi purtroppo noto, la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, alle ore 3,32, un fortissimo terremoto ha colpito l'Italia centrale e segnatamente la Regione Abruzzo, la città dell'Aquila suo capoluogo, e numerosi Comuni circostanti. Altissimo il tributo in vite umane (298 vittime), in feriti (oltre 1.500), in abitanti rimasti d'un tratto privi delle loro abitazioni (63.084). Rilevante il patrimonio immobiliare pubblico e privato distrutto o seriamente compromesso nella sua stabilità e integrità; profonda la ferita al patrimonio culturale, artistico ed architettonico del Paese che vede in quelle città concentrata alta e cospicua parte di sé. Altrettanto note a noi e al mondo sono l'immediatezza, la tempestività e l'efficienza con le quali le strutture della Repubblica, Protezione civile e Governo in testa, hanno spiegato i loro interventi di soccorso e di emergenza e tuttora svolgono la loro attività. *(Brusìo)*. Bastano le cifre:

Bastano le cifre: 33.964 persone alloggiate provvisoriamente in alberghi e case private nelle vicine province di Teramo, Pescara, Chieti e Ascoli Piceno; 29.120 persone alloggiate in 5.674 tende distribuite in 180 aree di ricovero; 103 cucine da campo; 35 presidi sanitari mobili; una cittadella delle istituzioni per consentire la provvisoria operatività di ben 38 uffici nazionali, regionali e provinciali presenti nella città dell'Aquila, e ulteriore, coerente numero di presidi ausiliari per attività scolastiche, sociali e così via; oltre 12.000 persone delle strutture pubbliche impegnate nell'opera di soccorso e di gestione dell'emergenza, in aggiunta ad un gran numero di volontari. Bastano le cifre - dicevo - per immaginare l'enorme sforzo organizzativo e di risorse che il Governo ha affrontato e affronta con grande impegno e determinazione, confortato dalla piena solidarietà della comunità nazionale e internazionale. Già alle ore 4 del mattino dello stesso 6 aprile l'unità di crisi della Protezione civile era riunita sotto la direzione del suo vertice, dottor Guido Bertolaso, Sottosegretario di Stato, e nel volgere di pochi minuti partivano dalla capitale le prime colonne di soccorso specializzato con in testa i nostri Vigili del fuoco. È grazie a tale tempestività ed efficienza se molte vite umane sono state salvate e molti feriti immediatamente ed utilmente soccorsi. Nella stessa giornata il Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi, firmava la prima ordinanza di protezione civile nella quale, oltre alle prime urgenti disposizioni, era contenuta la nomina dello stesso sottosegretario Bertolaso a commissario delegato per tutte le operazioni legate all'emergenza terremoto. Di tutte le successive ordinanze che hanno preceduto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, oggi al nostro esame, e di quelle che l'emergenza ha reso necessario emanare alla luce

il dettaglio analitico dell'oggetto dei singoli articoli del decreto del Governo. Riferirò piuttosto dei contenuti del dibattito svoltosi in 13a Commissione e delle principali modifiche a quel testo, che essa propone attraverso gli emendamenti approvati, anche su iniziativa del Governo. Procedo in tal modo perché ritengo preliminarmente doveroso doveroso dare risalto ai significativi aspetti innovativi, tanto di contesto normativo quanto di contenuti, adottati nella definizione delle fasi dell'intervento per l'emergenza Abruzzo.

trova nel decreto conferma al loro dettato e definizione di termini per quanto dei loro contenuti si ritiene debba permanere e per quelle in materia ancora da emanare. La seconda fase è quella dell'emergenza cosiddetta ordinaria. Si distingue per interventi connessi al bisogno primario e pressante del problema abitativo da risolversi in pochi mesi di tempo, prima che sopraggiunga l'inverno; il decreto ne disciplina gli indirizzi generali, gli ambiti soggettivi ed oggettivi, le coperture finanziarie. Per la sua stretta connessione con la fase della prima emergenza, ne individua ed autorizza nella stessa fattispecie dell'ordinanza lo strumento operativo, comprendendone anche l'eventuale necessario accavallarsi tra legge ed ordinanza in termini temporali, dovuto anche al progressivo aggiornarsi del quadro informativo proveniente dall'attività dei tecnici sul territorio.

fermo restando il principio assoluto del rispetto della gerarchia delle fonti normative e, quindi, del riallinearsi delle seconde, cioè delle ordinanze, ai contenuti della prima, cioè la legge, ove non siano con essa compatibili. La terza fase è quella della ricostruzione, elemento nuovo e qualificante dell'azione del Governo per l'immediatezza con la quale viene affrontata, nella volontà che l'Abruzzo non segua la sorte di altri territori nel passato interessati da analoghe tragiche vicende, e per la diffusa attenzione che riserva al contesto socio-economico produttivo, anche in questo caso con aspetti che legano la terza fase alla seconda per quanto attiene alcuni profili urbanistici e strutturali, ma anche con visioni di più ampio respiro oltre gli stessi confini che la norma territorialmente indica. Il decreto più puntualmente si sofferma sugli elementi soggettivi, sulla dimensione dei vari interventi, sui meccanismi finanziari che dovranno fare da rigorosa cornice ai contenuti delle ordinanze, che anche in questa fase trovano ragion d'essere perché funzionali a scopi di celerità ed efficienza e con caratteristiche di elevata discrezionalità da parte del Governo.

l'attenzione al territorio. È stato individuato, nella rilevazione fatta alla luce della scala Mercalli e precisamente del sesto grado della stessa, l'ambito territoriale al quale riferire alcune delle principali previsioni di questo decreto. Tale ambito è già stato identificato con una specifica ordinanza del Governo, che ha individuato in 49 Comuni

Questo è un dato oggettivo comune a tutte e tre le fasi dell'intervento. Naturalmente vi è la possibilità che, man mano che procedono le rilevazioni, il commissario delegato rilevi che vi sono altri territori che hanno subito la stessa intensità media del danno e che quindi possono essere aggiunti a quell'elenco. Gli elementi soggettivi sono principalmente gli abitanti. Nella prima fase, chiunque si trovasse nel luogo del disastro al momento del suo verificarsi è stato adeguatamente ed immediatamente oggetto dell'assistenza predisposta. Nella seconda fase, quella dell'apprestamento e del reperimento delle unità abitative prima dell'inverno,

un diverso trattamento tra beni destinati ad abitazione principale ed altri beni abitativi, affermandosi, per quelli destinati ad abitazione principale, il principio dell'intera ricostruzione e dell'intero risarcimento del danno, anche se non letale. Si passa poi a trattare della ricostruzione degli edifici pubblici, delle strutture produttive, dei beni culturali, con una particolare attenzione per i centri storici, attraverso una serie di modalità di intervento. Sulle strutture produttive, la Commissione ha rilevato che occorre intervenire anche per quanto riguarda l'attività

abbiamo individuato tre essenziali momenti. Il principale è quello della costruzione di moduli abitativi che abbiano una loro valenza strutturale, duratura nel tempo, in modo da mettere in grado i loro abitanti non solo di affrontare

A questi si accostano gli alloggi reperiti sul territorio, che sono numerosi, per quello che ci riferiscono i tecnici occupati nella rilevazione e il reperimento,

al momento dell'assegnazione dei moduli abitativi o degli stessi alloggi avranno ancora la necessità di un'utile sistemazione. La Commissione ha ulteriormente aggiunto un emendamento relativo alle piccole riparazioni con l'intento preciso di intervenire su quelle abitazioni che con poco intervento possono essere ripristinate e che quindi possono diminuire il carico per la costruzione dei nuovi moduli abitativi o per l'affitto degli alloggi da reperirsi e possono anche assolvere ad uno scopo che in tutto il dibattito in Commissione è stato ritenuto uno degli degli obiettivi principali da perseguire, quello cioè del mantenimento della coesione sociale della comunità abruzzese, segnatamente della città dell'Aquila. È infatti la prima volta, signor Presidente, che un terremoto, dopo quello disastroso

capoluogo di Regione, con la presenza, come dicevo poco fa, di ben 38 uffici pubblici finalizzati all'assolvimento di tale ruolo. Questo è stato quindi uno degli elementi che hanno contraddistinto il dibattito in Commissione. Tutti abbiamo riconosciuto la necessità di mantenere alla città dell'Aquila, anche se in condizioni precarie, il suo ruolo operativo

rivolgono alle istituzioni perché non si disperda questo coeso tessuto sociale, accontentandosi di vivere i momenti di transizione anche in stato di disagio pur di non perdere tale compattezza.

stabilisce che lo Stato si accolli, nella misura massima di 150.000 euro, anche i mutui in essere per la costruzione dell'abitazione principale. Ciò in aggiunta, signor Presidente e colleghi, al provvedimento

alla ricerca della loro prima abitazione, si erano gravati di un finanziamento pluriennale. È stata anche chiarita la possibilità dell'utilizzo del credito d'imposta, che si avrà solamente su base volontaria, e forse il dibattito in Aula potrà potrà chiarire ulteriormente le modalità con cui, attraverso le ordinanze, si potrà poi procedere all'utilizzo dello stesso credito di imposta per il pagamento, per chi lo volesse, di eventuali finanziamenti agevolati posti in essere in vece di contributi diretti.

le analisi degli eventuali danni e la necessità di eventuali immediati interventi per mettere in sicurezza tutte le infrastrutture che quotidianamente presiedono alle esigenze dei trasporti in quella zona.

importanza il ruolo del Presidente della Regione, che viene costantemente affiancato a quello del commissario delegato.

ma su indicazione di tutti i componenti della Commissione - per l'istituzione di una zona franca urbana nel territorio della Provincia dell'Aquila. Su questo punto il Governo ha convenuto ed ha stanziato le risorse necessarie. Immagino altresì che l'Esecutivo abbia già attivato le procedure autorizzative indispensabili in sede comunitaria perché la zona franca urbana possa essere uno degli strumenti fondamentali affinché il territorio abruzzese, e segnatamente quello della Provincia dell'Aquila, possa rapidamente riprendere la sua corsa verso lo sviluppo economico e sociale.

prodotti dai crolli o dalle demolizioni che si renderanno indispensabili. Come ho ricordato inizialmente, la norma affronta con più ampio respiro anche tematiche di rilievo nazionale o di protezione civile nella sua Tutta la Commissione ha sottolineato e condiviso l'importanza dell'articolo 11 ed ha introdotto alcune modifiche ritenute utili per meglio applicarlo sull'intero territorio nazionale. nazionale. La Commissione ha inoltre convenuto sull'emendamento del Governo per quanto riguarda l'attenzione particolare per i centri storici.

finanziario del Governo, che dovrà intervenire in questa fase della ricostruzione. Signor Presidente, volendo adesso

la tempestività con la quale tale provvedimento è stato assunto dal Governo; a ciò si accompagna la tempestività nell'intervento operativo e quindi l'assistenza immediata alle popolazioni vittime del sisma.

cioè per la fase dell'immediata emergenza e per quella che ci costringe ad una tempestività assoluta nell'apprestamento delle abitazioni provvisorie

tratta di un atto, come dicevo, di assunzione di responsabilità, perché la sfida è assolutamente importante ed è anche non dico difficile, perché non voglio creare dubbi sul suo esito, ma estremamente impegnativa:

confortevole, ma certamente transitoria, e di farlo entro l'arrivo dell'inverno; una sfida che il Governo si è assunto nelle sue dirette responsabilità e che noi non possiamo,

è forte, ma minare con il presupposto, anche solamente teorico, che vi possano essere poteri interdittivi alle decisioni urgenti e fondamentali che presiedono questo percorso.

più volte criticata anche dall'opposizione, di «sentiti» piuttosto che non «d'intesa»: di fatto diventa un'intesa, ma dal punto di vista formale la *governance* in questa fase - ripeto - non può che essere rimessa all'intera responsabilità

sul coinvolgimento, anche formale (ciò è dimostrato anche dal contenuto degli emendamenti presentati dallo stesso Governo), dei livelli locali per tale passaggio. un quadro che, come si sono permesso di segnalare all'inizio, può e deve subire anche modifiche perché stiamo intervenendo solamente a poco più di un mese; lo stesso decreto-legge interviene ancor prima della scadenza dei 30 giorni dall'avverarsi dell'evento calamitoso. Si tratta di un quadro che può e deve aggiornarsi a seguito delle costanti e continue rilevazioni che gli organi tecnici stanno compiendo sul territorio. Ad esempio, sappiamo che oltre il 50 per cento delle abitazioni che sono già state sottoposte a verifica è stato dichiarato agibile e, quindi, oltre il 50 per cento dei 62.000 abitanti attualmente e provvisoriamente collocati in altre strutture potrà potrà rientrare nelle proprie abitazioni anche a seguito di piccoli interventi di manutenzione; così pure sappiamo che questo numero potrebbe sensibilmente crescere. Pertanto, alla fine, la costruzione dei nuovi moduli abitativi potrà interessare un numero

Signor Presidente, credo che dal punto di vista della tensione emotiva ma anche della collaborazione politica questo provvedimento sia stato affrontato in Commissione con animo assolutamente sereno da tutti i suoi componenti. Lo stesso spero che possa accadere in Aula, così come spero che, al di là di ogni polemica che potrebbe oggi

Stiamo infatti lavorando tutti insieme nell'interesse di una popolazione che ci è vicina e che è stata colpita da un evento calamitoso di proporzioni veramente straordinarie.

e non dall'altra.

nella fase della prima emergenza dopo il terremoto del 6 aprile, come di fronte a questo decreto che deve gettare le basi per la ricostruzione, il Partito Democratico ha mostrato intenzioni e disponibilità di piena collaborazione, come del resto era nostro dovere in un caso nel quale l'abituale dialettica tra maggioranza e opposizione deve fare più di un passo indietro e invece deve prevalere uno sforzo unanime di solidarietà nell'aiuto a chi ha sofferto e soffre per le conseguenze di una grande tragedia nazionale

In questo decreto, però, noi, come gran parte degli amministratori, delle forze economiche e sociali, dei cittadini dell'area colpita dal sisma, abbiamo segnalato da subito almeno due grandi equivoci. Il primo equivoco era nella vaghezza della garanzia a chi ha avuto beni immobili, in particolare la casa d'abitazione, distrutti o danneggiati di vedersi riconosciuto il diritto a un'integrale copertura delle spese necessarie a ricostruire o a riparare. ricordo, che è stato costantemente affermato in tutti i casi precedenti della nostra storia più o meno recente. Nel testo del decreto oggi in vigore questo diritto non c'era, come non c'era una chiara indicazione delle risorse necessarie per finanziare la ricostruzione. Grazie alle proposte e alla pressione del Partito Democratico, delle altre opposizioni e degli amministratori abruzzesi, le modifiche apportate al decreto in Commissione hanno dato una prima, importante risposta alle legittime preoccupazioni dei cittadini dell'Aquila e degli altri Comuni colpiti dal sisma, specialmente per ciò che riguarda le case di abitazione principale. Ma come diranno meglio di me altri colleghi, restano incertezze sulle coperture finanziarie in particolare per l'anno in corso resta largamente imprecisato - nei tempi, nelle modalità, nell'entità - il sostegno alla ripresa delle attività produttive, di servizi e professionali, e alla ricostruzione delle case non di abitazione principale, che costituiscono una parte rilevante del patrimonio distrutto o gravemente danneggiato, specialmente nei centri storici e agli interventi nei Comuni esterni al cosiddetto cratere, ma che hanno comunque subito danni rilevanti. Il secondo equivoco di questo decreto, ad oggi sostanzialmente irrisolto, è nel fatto di estendere l'affidamento esclusivo al commissario delegato delle funzioni di gestione dell'emergenza ben al di là della fase del primo soccorso. l'idea del Governo è che, non per alcuni mesi, ma per i prossimi anni, la gran parte delle funzioni di governo nei territori colpiti dal sisma sarà nelle mani di un'istituzione monocratica qual è il commissario. Per quanto possa essere grande la stima e la considerazione per il sottosegretario Guido Bertolaso, che ad oggi è titolare di tale funzione, noi riteniamo questa scelta un grave errore. Faccio un esempio concreto per chiarire il senso della nostra posizione. È stato deciso di realizzare in tempi brevissimi, entro l'inizio dell'autunno (come hanno più volte dichiarato il sottosegretario Bertolaso e lo stesso Presidente del Consiglio), aree con i cosiddetti moduli, dove abiteranno stabilmente 15.000 persone per il tempo necessario a vedere ricostruite o riparate le loro case. Naturalmente l'obiettivo in sé è lodevole e condivisibile, a patto che i tempi siano rispettati alla lettera, visto che in ottobre all'Aquila farà già molto freddo. Ma questa scelta comporta conseguenze importanti: di fatto, vuol dire che si comincia subito la ricostruzione. Infatti, le aree con i moduli non rimarranno lì solo per qualche anno, ma resteranno per sempre: si tratta di una zona di circa un chilometro quadrato (se la densità è quella dichiarata in Commissione dal sottosegretario Bertolaso), che cambierà in modo definitivo il volto urbanistico dell'Aquila e degli altri Comuni coinvolti. ma una simile scelta, che già riguarda squisitamente la ricostruzione, non può essere soltanto nelle mani del commissario, non può passare sopra le competenze ordinarie delle istituzioni del territorio, prime fra tutte i sindaci. La localizzazione delle aree, in base al testo del decreto-legge, viene fatta senza il parere vincolante dei sindaci, senza garanzie di qualità e coerenza urbanistica e addirittura, secondo un emendamento della maggioranza approvato in Commissione, prevedendo espressamente la deroga alle norme igienico-sanitarie (come se si trattasse di strutture provvisorie, non definitive). Insomma, nascerà una L'Aquila parallela, fatta di tante piccole *new town*, e io penso che le comunità locali non possano essere solo spettatrici di questa fase; altrimenti per la prima volta un pezzo di città legale nascerebbe per ordinanza di un'autorità monocratica, fuori da ogni controllo democratico e anche, aggiungo, in aperto contrasto con ripetute sentenze della Consulta (l'ultima nel 2005) che individuano nei Comuni i titolari esclusivi degli strumenti urbanistici attuativi. Il commissario può e deve gestire la prima emergenza con la massima rapidità d'intervento, ma la ricostruzione deve vedere protagonisti, e non semplici attendenti generosamente tenuti informati delle decisioni, coloro ai quali i cittadini hanno affidato la loro fiducia. Con questo schema di decreto, per la parte riguardante la *governance*, la conseguenza sarebbe invece che per alcuni anni in una parte di territorio italiano verrebbero sospese le garanzie democratiche relativamente a scelte importanti. Chiudo su un tema che personalmente mi sta molto a cuore, rappresentato dalle verifiche antisismiche, uno dei punti più innovativi del testo in esame, che prevede, a partire dalle zone contigue a quelle colpite dal terremoto, l'avvio di un programma di controlli su tutte le abitazioni finalizzato ad accrescerne la sicurezza antisismica. Nel decreto approvato dal Governo mancavano al riguardo due punti importanti: l'attivazione immediata delle norme antisismiche per tutte le nuove costruzioni, introdotte nel 2004 ma poi ripetutamente prorogate, e l'inclusione dei lavori di adeguamento antisismico tra gli interventi per i quali è prevista la detraibilità fiscale del 55 per cento La prima lacuna è stata colmata in Commissione con l'accoglimento degli emendamenti presentati dai Gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori; sulla seconda ci aspettiamo che in Aula si possa arrivare ad una soluzione positiva, tanto più urgente visto che sembra sia slittato ad agosto il piano casa che avrebbe dovuto contenere entrambe le norme.

onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, pensare che nel nostro Paese gli eventi sismici e, più in generale, gli eventi calamitosi siano un'eccezione, costituisce un grave errore. Terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, venti sciroccali

pronta e professionale, come quella di cui l'Italia dispone e per la quale ha ottenuto l'apprezzamento di tutti in più occasioni. Ma proprio perché le calamità naturali non costituiscono un'eccezione, è necessario fare tesoro delle esperienze sin qui maturate, facendo sì che le stesse rappresentino un modo utile per implementare l'attività di protezione civile, migliorandone i risultati. È di tutta evidenza, onorevoli colleghi, che le fattispecie a cui far fronte in occasione di un evento calamitoso sono il più delle volte standard. Mi riferisco ai soccorsi, all'emergenza, all'assistenza, ma pure alla ricostruzione, ai danni e al loro risarcimento. Anche l'evento sismico che ha colpito l'Abruzzo, e che ha prodotto un'ondata di solidarietà straordinaria ed entusiasmante in tutto il mondo, deve costituire l'occasione per migliorare le capacità di intervento della nostra protezione civile e, più in generale, le capacità di intervento del Governo in casi del genere. Le parole chiave a cui dobbiamo pensare sono: tempestività, organizzazione, professionalità, solidarietà, sinergia, prevenzione, vigilanza, controllo. Tutte questioni a cui la legge che stiamo discutendo offre una soluzione che non può e non deve costituire un intervento buono solo per questa drammatica circostanza, come non lo sono state, sia sia pure in parte, quelle adottate in precedenza per l'Irpinia, per il Vajont, per il Belice, per l'Etna, per Siracusa ed altri eventi del passato. Intendo dire che le problematiche che si ripropongono non possono essere considerate straordinarie, né straordinarie possono essere considerate le soluzioni che vengono adottate. Il Governo, con questo provvedimento, compie un notevole passo in avanti, ma è venuto il momento per fare di più,

il varo di un provvedimento organico che, per una volta, non sia il frutto della tragica contingenza degli eventi ma dell'esperienza che gli eventi stessi hanno determinato da parte della nostra Protezione civile e del nostro Governo nel tempo. Mi riferisco, intanto, ad un organico stabile di personale specializzato, sia nelle funzioni centrali, come già accade, sia nei territori ed in particolare nei Comuni e nelle Regioni. Se gli eventi calamitosi, purtroppo, non costituiscono un'eccezione, non possono costituire un'eccezione le politiche che devono essere poste in essere per la loro prevenzione e per gli interventi ad essi, di volta in volta, conseguenti. In Sicilia quasi l'intero organico, peraltro esiguo, della Protezione civile è in servizio in virtù di contratti a termine, mentre a termine non possono essere, né la prevenzione, né l'azione di protezione civile, in quanto costanti sono le calamità a cui far fronte. I fondi per le politiche di prevenzione, per le politiche della ricostruzione, per le politiche della casa, per le politiche della ripresa sociale ed imprenditoriale non possono essere disposti di volta in volta. Essi devono costituire una costante del bilancio dello Stato, così come una costante deve essere l'assetto normativo di riferimento riguardante gli aiuti alle persone, alle famiglie ed alle imprese. Penso ad una legge quadro sulla Protezione civile che disciplini la prevenzione, il personale, gli aiuti, il volontariato, la ricostruzione, il controllo e la ripresa economica, a cui far riferimento non di volta in volta, bensì sempre e sempre con le e sempre con le risorse necessarie, anche attraverso il supporto di sistemi assicurativi chiari ed adeguati, capaci di integrare i necessari fondi pubblici e quelli frutto della generosità degli italiani e non solo degli italiani. La legge che stiamo discutendo - e concludo, onorevoli colleghi - risponde in parte a queste esigenze e costituisce un ulteriore tassello di quel mosaico che deve rappresentare la protezione civile italiana. Ma guai a fermarsi, guai a non anticipare i tempi, guai a pensare che anche questo terribile terremoto dell'Abruzzo costituisca un'eccezione. Esso è parte di una costante del nostro territorio e come una costante deve essere affrontato. So che il Governo saprà fare il suo dovere e so pure che lo farà in fretta e con competenza, soprattutto se il Parlamento saprà comprendere che, su fenomeni drammatici di questo tipo, non ci si può dividere, anzi bisogna marciare compatti e con grande velocità, come compatta e tempestiva è stata, fino ad oggi, la solidarietà di tutto il Paese

Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, in merito alla tragedia che ha colpito l'Abruzzo, maggioranza ed opposizione avrebbero il dovere di trovare le più ampie convergenze per offrire risposte serie ed unitarie ai cittadini colpiti dal sisma. Tuttavia non è facile evitare la polemica rispetto ad un decreto che, almeno nella sua prima stesura, non aveva preventivato alcun tangibile aiuto economico per la ricostruzione, salvo proventi aleatori, 500 milioni di euro, derivanti da lotto e lotterie, prevedendo al contrario, come è prassi di questo Governo, argomenti estranei come il riordino del Ministero dell'economia. Da senatori abruzzesi abbiamo seguito la disgrazia sin dai primi giorni, fatto la spola con le zone colpite e, su segnalazione dei medici del San Salvatore,

A distanza di 40 giorni il quotidiano "la Repubblica" di ieri denuncia la situazione insostenibile di quell'ospedale: un tendone militare con dentro 27 malati, un letto dietro l'altro, circondato da fango, detriti, erbacce, liquami e rifiuti; pochi metri più avanti, cinque bagni chimici all'aperto "riservati ai malati" o almeno a quei pochi di loro che riescono ad alzarsi: eccolo qui il reparto di medicina interna dell'ospedale da campo San Salvatore! Ecco i posti letto! Come hanno denunciato Vittorio Festuccia (primario di medicina generale), Sabrina Cicogna (cardiologia) e Giovanni Flati (dermatologia), «è impossibile continuare in queste condizioni»; all'ospedale da campo c'è una «situazione di promiscuità e scarsa igiene» che, favorita dal caldo intenso, «condiziona il diffondersi di malattie batteriche». «Occorre intervenire subito. Bisogna immediatamente attivare l'ospedale da campo del G8, come era stato annunciato diverse settimane fa». E concludono amaramente: «Molti a parole si dicono impegnati nel mantenimento di una città di livello per ogni settore, sanità, istruzione, lavoro e qualità complessiva della vita, pochi in realtà sono stati realmente fattivi e utili al raggiungimento dello scopo». Accogliendo alcune richieste delle opposizioni, il Governo e il relatore hanno accettato di modificare alcuni parti del decreto-legge per stabilire che il contributo dello Stato per le prime case distrutte, inagibili o anche danneggiate dal terremoto del 6 aprile sarà tale da coprire integralmente le spese per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. Vengono in tal modo accolti tre rilievi dell'Italia dei Valori, cui corrispondevano altrettanti emendamenti: l'estensione dei contributi anche alla case danneggiate, la copertura al 100 per cento dei danni e la specificazione che il contributo viene erogato a fondo perduto. La debolezza del decreto è rappresentata però dalla mancata indicazione, nero su bianco, delle somme che saranno messe a disposizione dei cittadini e dei Comuni per l'immediata ricostruzione. Di fatto, sono indicate con precisione solo le risorse per le casette transitorie. Un primo punto da correggere, per evitare problemi nell'azione di ricostruzione, è quello relativo all'eccessivo accentramento (come sottolineato anche da chi mi ha preceduto) dei poteri decisori e autorizzatori nelle mani del Governo centrale, che opera tramite il commissario delegato, dopo aver semplicemente «sentito gli enti locali». Noi abbiamo stima, come tutti quanti, del commissario straordinario, però non si può mettere tutto nelle mani di un solo uomo che, come tutti gli uomini, può essere fallibile. A fronte di interventi così complessi e prolungati nel tempo, tale impostazione andrebbe trasformata in un'intesa con gli enti locali, anche perché tale via è stata seguita per Marche, Umbria e Friuli. Quanti si trovano a dover pagare un mutuo sulla casa distrutta, purché non morosi, a parte la sospensione prevista in termini generici, avranno la possibilità di vedere il subentro dello Stato nel debito contratto con le banche,

subentra per l'importo del contributo dal quale si detrae il prezzo ricevuto da Fintecna, mentre al proprietario resterebbe parte del contributo previsto ed un eventuale nuovo mutuo da stipulare. Gran parte degli 8,5 miliardi di euro annunciati (ammontante però a poco meno di 6 miliardi) sarà disponibile solo in un arco di tempo di 24 anni. Per il primo biennio sono stanziati effettivamente 1,7 miliardi con riferimento a tale biennio, per le case di transizione si prevedono risorse anche nel 2010, con il rischio, quindi, che esse non siano ultimate entro la fine dell'estate, come promesso. E chi vive in Abruzzo, o è abruzzese, sa è abruzzese, sa che a L'Aquila l'inverno comincia dai primi di ottobre, ed è un inverno terribile. Nel complesso, poco meno del 60 per cento delle risorse è rimesso ad entrate virtuali o ipotetiche (giochi, lotterie, che coprono circa 4,5 miliardi dell'importo), condizionate da eventi futuri ed aleatori. Mancano riferimenti chiari e puntuali ai contributi a fondo perduto per la ricostruzione e la riparazione. Parte della copertura è realizzata attraverso l'utilizzo dei fondi destinati al *bonus* per le famiglie bisognose ed una diversa modulazione del fondo FAS che, come tutti sappiamo, è già stato saccheggiato dal Governo a copertura di altri provvedimenti. Mancano indicazioni chiare sulle procedure e sull'entità dei contributi destinati alla ricostruzione degli immobili industriali e commerciali danneggiati. Non sono chiari i tempi di erogazione, né l'importo massimo; anche in questo caso non si tratterà, in gran parte, di soldi liquidi, bensì di finanziamenti indiretti attraverso il meccanismo del credito d'imposta, in una zona dove la capacità reddituale potrebbe scendere notevolmente, almeno nell'immediato. Non è disciplinata, per le aziende che avessero necessità di accelerare i tempi della burocrazia, la possibilità di ricorrere a perizie

scritto: «A me pare di estrema gravità che in questo momento si blocchi uno strumento di pagamento persone in stato di difficoltà, solo per il dubbio che, essendo terremotati, possano diventare insolventi, dubbio che nel mio caso particolare è poi insussistente, essendo io un pubblico dipendente». Signor Presidente, noi

La prima riguarda l'eccezionalità di questo evento tragico,

è capoluogo di Regione. Si è creata, quindi, una sorta di buco nero nel centro di una Regione e nel centro dell'Italia, che occorre al più presto

trascorso dal terremoto. Il secondo dato, signor Presidente, colleghi, è quello della originalità, della particolarità del provvedimento governativo, non solo perché interviene a soli venti giorni dall'evento sismico,

lasciarsi andare ritenendo che la loro vita non possa mai tornare quella che è stata fino alla notte tra il 5 e il 6 aprile di quest'anno. Questo pregio del decreto‑legge deve essere valutato, apprezzato e considerato nel suo giusto rilievo. È chiaro che viviamo una situazione ancora sfumata, non definita in tutti i suoi dettagli: proprio perché il provvedimento immediato ha voluto metter mano e provvedere a queste due emergenze allo stesso modo, vi sono dei punti che sono soggetti ad essere rivalutati e riconsiderati. Da qui nasce

sul territorio potrà intervenire in un modo piuttosto che in un altro. Questo decreto, però, contiene dei punti fermi: sappiamo che nelle Commissioni, anche in quelle che hanno rilasciato dei pareri (compresa quella di cui faccio parte

non si riferisce a spese da effettuarsi nel 2032, bensì alla spalmatura del debito che può arrivare fino a quell'anno, ma per spese che vengono effettuate nei tempi e nei modi previsti dal decreto-legge, che ci auguriamo siano tempi strettissimi e modi assolutamente soddisfacenti. Ciò è tanto vero che dal dibattito e dal confronto nella Commissione di merito sulla copertura non vi sono state modifiche né riformulazioni, se non su alcune questioni di dettaglio. secondo punto è quello relativo alla definitività o meno del decreto del Commissario delegato all'individuazione dei Comuni colpiti in maniera più rilevante, quelli che appartengono al cosiddetto cratere, alla parte attraversata in maniera più diretta dal terremoto. Credo che il provvedimento - come tutti - non sia definitivo, ma che le

futuro: sarà ancora più definitivo quanto meglio saranno stati valutati questi elementi. È stato fatto riferimento a quel livello della scala Mercalli (il sesto grado) che ha dei parametri ben precisi.

spero si possa intervenire in fase emendativa - che sarebbe eccessivamente estensibile al di fuori dei Comuni colpiti in maniera più violenta Un'altra questione che ha appassionato i lavori della 13a Commissione e della Commissione affari costituzionali, perché poneva problemi di graduazione degli interventi, è stato quello sulla ricostruzione.

prevedendo la copertura dei danni o della ricostruzione integrale al cento per cento del costo: mi sembra che ciò rappresenti un passo decisamente importante per dare maggior tranquillità e sicurezza ai cittadini aquilani che hanno subito un *vulnus* così profondo. Un'ultima questione, colleghi, è stata quella delle deroghe al sistema delle competenze istituzionali degli enti territoriali.

che un commissario delegato o un'autorità governativa potesse intervenire in materia urbanistica o edilizia per modificare regolamenti o piani regolatori. Non è scritto da nessuna parte ed è chiaro che quelle autonomie sono conservate e vanno

che ogni istituzione ha le sue responsabilità, i suoi ruoli e il suo campo d'azione. Non possiamo pensare che istituzioni che provvedono solo ad aspetti particolari particolari della gestione pubblica possano, a causa del terremoto, assurgere a soggetti quasi sovraordinati rispetto ad altri, e mi riferisco

siano state date risposte alle perplessità che sono state espresse in questi giorni di dibattito e che il provvedimento esca dalla Commissione molto migliorato. Vi sono ancora alcuni passaggi da precisare.

Al di là di questi dati puntuali, il provvedimento oggi è senz'altro più che soddisfacente. È un provvedimento che dà una risposta concreta all'emergenza di oggi e soprattutto

le forze dell'ordine, la Protezione civile, i volontari, i Vigili del fuoco, l'Esercito e quanti si sono prodigati ad alleviare le sofferenze e a prestare i primi soccorsi al popolo abruzzese colpito dal violento sisma del 6 aprile scorso. La prontezza dei soccorsi, guidati con perizia e grande capacità dal sottosegretario Bertolaso e la presenza del Governo fin dalle prime ore della tragedia hanno consentito di dare immediate e concrete risposte all'emergenza, oltre che testimoniare la presenza dello Stato con, in testa, il Presidente del Consiglio, che infaticabilmente ha presenziato alle attività di coordinamento e di prima emergenza e che ha, nei giorni successivi, con dieci ordinanze e, in modo particolare, con il decreto‑legge oggi dato risposte e prospettive di ricostruzione delle unità abitative, di quelle produttive, ma soprattutto di quelle socio-economiche.

e collaborativo lavoro svolto dalla Commissione di merito. Si tratta di un provvedimento che ritengo di particolare importanza e che apre, oltre alla ricostruzione dei nuclei abitativi a totale carico dello Stato, così come è chiarito da un emendamento che smentisce una campagna disinformativa messa in campo in questi giorni, anche ad una prospettiva di ripresa dopo il terremoto. Voglio subito dire che la prima questione che abbiamo affrontato, ancora prima della Commissione di merito, è stata

l'anno. La copertura maggiore è al comma 1 dell'articolo 14 a valere sul Fondo strategico per le aree sottoutilizzate, copertura che è stata accertata con Nota del Ragioniere generale dello Stato. Stato. Con queste coperture finanziarie si dà attuazione al piano per le 20 aree abitative che, una una volta ricostruite le abitazioni, potranno essere messe a disposizione degli studenti universitari: si tratta di un progetto di costruzione di circa 6.000 moduli abitativi per 15.000 persone. Per questo esiste una copertura finanziaria ben precisa, sempre a valere al comma 1 dell'articolo 14 e che stima in 700 milioni di euro la costruzione di questi moduli per 15.000 persone. È una scelta coraggiosa, che tende a sistemare entro l'inverno le sicuri, vere e proprie case, anche se transitorie, che poi rimarranno comunque nella dotazione del patrimonio dell'edificato del Comune dell'Aquila e dei Comuni limitrofi.

riguardano l'emergenza sanitaria, l'emergenza abitativa (con quei fondi si pagheranno gli indennizzi per gli alberghi e le abitazioni private messe a disposizione

Il decreto in esame promuove anche una piccola rivoluzione culturale, quando definisce con precisione l'elenco dei Comuni interessati, le linee portanti e gli obiettivi fondamentali dell'intervento statale, non solo di prima emergenza. L'elenco dei Comuni interessati è stato un altro oggetto delle polemiche di questi giorni, polemiche comprensibili, perché sindaci e popolazioni di Comuni che comunque hanno subito danni e che si trovano oggi al di fuori del cosiddetto cratere, cioè dei 49 Comuni compresi nel decreto di Protezione civile del 16 aprile, naturalmente hanno ritenuto di essere stati abbandonati delle provvidenze per la ricostruzione e la riparazione anche degli edifici pubblici dei loro territori. Credo che il comma 3 dell'articolo 1 chiarisca tale aspetto

avuto e non hanno bisogno di interventi per l'immediata emergenza, avranno bisogno di interventi legati al discorso ricostruzione ed il comma 3 dell'articolo 1 copre anche questo tipo di esigenze nelle zone al di fuori del cratere individuato dal decreto di Protezione civile del 16 aprile scorso. innovazioni degli emendamenti approvati in Commissione è costituita dalla zona franca urbana per la Provincia dell'Aquila, su cui naturalmente si dovrà aspettare un *placet* europeo,

e dovrà anche stabilire i criteri di assegnazione. Per questo, il Fondo previsto nella finanziaria 2007 per le zone franche urbane, di 50 milioni di euro per il 2009, è stato incrementato di 45 milioni di euro, che costituiscono

a chi ha capienza di reddito di richiedere una parte di risarcimento a fondo perduto, immediata, e una parte di risarcimento con credito d'imposta. È chiaro che, con la possibilità

da sistemare nei moduli provvisori. Ritengo quindi che il testo di quell'emendamento vada portato al di fuori dell'articolo 2, magari

del 2002. Mi preme innanzitutto esprimere grandissima solidarietà umana al popolo abruzzese, a quelle comunità che hanno subito una delle più grandi tragedie che possano capitare ad un popolo.

convinto di questo: si rispetta il popolo abruzzese, si rispetta chi ha subito questi gravi danni con la presenza in Aula, dibattendo insieme a noi su quello che bisogna fare.

i diritti vanno stabiliti per legge. Nei prossimi giorni presenterò, in base alla mia esperienza, una modifica a questa

le disgrazie debbano avere una risposta uguale per tutti, in tutta Italia. Ecco perché i diritti delle persone devono essere fissati per legge.

Sulla sofferenza, sul bisogno, sulla ricostruzione non devono esistere strumentalizzazioni sottili, anche di ordine politico. Al

che ancora una volta ha portato davanti agli occhi di tutti la tempestività dell'intervento del Governo, la tempestività della macchina dei soccorsi coordinata dal sottosegretario Guido Bertolaso, che si è mossa con grande rapidità per affrontare l'emergenza, ma anche la grande forza del del volontariato, che ancora una volta ha dimostrato come la cultura della solidarietà sia forte nel nostro Paese. Il compito della politica deve allora essere anche quello di valorizzare queste esperienze, favorendo il principio di sussidiarietà. è proprio dall'esigenza di fronteggiare l'emergenza e di avviare al più presto la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma, che nasce il provvedimento oggi al nostro esame. La parte pregnante è rivolta a prevedere una serie di interventi a favore dei territori e degli enti locali abruzzesi interessati dal terremoto: dalla realizzazione urgente di abitazioni, alle agevolazioni per la ricostruzione, dagli indennizzi a favore delle imprese, alla ricostruzione degli uffici pubblici. Per questo fine l'articolo 5 prevede, per esempio, la sospensione fino al 31 luglio 2009 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti alla data del sisma presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei Comuni colpiti dal sisma. Per questo è stata prevista per la ricostruzione di abitazioni principali distrutte o inagibili o per l'acquisto di abitazioni sostitutive la concessione di contributi, anche con il sistema del credito d'imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato; per le abitazioni non principali, contributi anche in credito d'imposta; in favore di attività produttive, indennizzi per la riparazione e ricostruzione degli immobili distrutti e inagibili. L'articolo L'articolo 10 contiene una serie di disposizioni volte ad agevolare lo sviluppo economico e sociale. In particolare, viene costituito un fondo di garanzia per la concessione di garanzie a titolo gratuito per i crediti bancari a piccole e medie imprese e studi professionali che insistono sulle zone colpite dal terremoto. Si dispone, inoltre, l'esenzione da costi e tributi, con eccezione dell'IVA, e così anche, per esempio, la riduzione del 50 per cento degli onorari notarili per le operazioni di rinegoziazione dei mutui. Si prevedono anche degli interventi per i giovani, si destina alla Regione Abruzzo una quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili, per le iniziative dirette alle giovani generazioni dell'Abruzzo. Così come si autorizza, per quanto riguarda le pari opportunità, la spesa di 3 milioni di euro per il 2009 a valere sul Fondo per le pari opportunità, a sostegno degli oneri di ricostruzione, restauro di immobili situati nei Comuni indicati all'articolo 1 e adibiti ad attività di centri di accoglienza, ascolto e aiuto a donne e madri in situazioni di difficoltà. E poi c'è l'intervento della Cassa depositi e prestiti, che storicamente finanzia gli investimenti degli enti locali attingendo al risparmio postale, che nel corso degli anni ha assunto una funzione sempre più rilevante nel finanziamento delle grandi opere infrastrutturali e e nella gestione della partecipazione dello Stato alle aziende pubbliche. Viene disposto che la Cassa depositi e prestiti proceda con una serie di interventi a favore delle popolazioni colpite colpite dal terremoto, a partire dalla sospensione delle rate dei mutui per un anno e dalla rinegoziazione degli stessi mutui con i Comuni. Secondo la relazione tecnica al decreto-legge il credito di imposta necessario per ricostruire il patrimonio edilizio privato danneggiato o distrutto dal terremoto è stimato in 3,162 miliardi di euro. Ma è prevista tutta una serie di altri interventi. Per esempio, ai privati obbligati alle verifiche edilizie per la riduzione del rischio sismico è riconosciuto un credito d'imposta del 55 per cento. Inoltre, la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione sarà di sei mesi: i destinatari del provvedimento sono 3.800, con un impatto sui conti dell'INPS pari a 23 milioni di euro nel 2009 e 30 milioni I lavoratori autonomi che potrebbero aver subito danni all'attività sono stimati in 11.700; per loro sarà prevista un'indennità di 800 euro mensili per un massimo di tre mensilità. Sarà quindi ingente l'impegno che dovrà essere sostenuto dall'erario. Per questo, come ha specificato il sottosegretario Giorgetti intervenendo in Commissione finanze, la scelta del Governo di reperire le risorse da destinare alla ricostruzione nella Regione Abruzzo, senza intervenire sul versante della spesa pubblica, risponde all'esigenza di tenere conto dell'attuale quadro congiunturale, sia macroeconomico, che di finanza pubblica. È quindi appropriata anche la copertura finanziaria individuata attraverso le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'offerta dei giochi con le disposizioni previste dall'articolo 12. Bisogna, infatti, sottolineare che si tratta di un meccanismo di contribuzione su base volontaria. Di qui, dunque, la scelta del Governo di inserire nel decreto-legge un corposo intervento sul settore dei giochi, tenendo però sempre presente l'impegno, assunto dallo stesso Esecutivo e ricordato dal sottosegretario Giorgetti, di presentare al Parlamento un'organica proposta di riforma dell'intero settore, che tenga conto di tematiche specifiche come i controlli, il quadro sanzionatorio e le misure di contrasto alla dipendenza. A questo fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può porre in essere, in base all'articolo 12, con propri decreti, una serie di misure finalizzata al reperimento di maggiori entrate, complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno in corso: previsione di entrata sottostimata rispetto all'andamento del settore, sempre secondo quanto ha sostenuto il sottosegretario Giorgetti. Si prevedono inoltre misure organizzative dirette ad incrementare l'azione di contrasto all'evasione fiscale attraverso una maggiore attività di controllo sul territorio. L'articolo 14 stabilisce che le maggiori entrate che provengono dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, siano assegnate ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, che sarà destinato sempre a misure in favore della popolazione colpita Infine, per concludere, dobbiamo ricordare che l'Italia è un Paese ad elevato rischio sismico e idrogeologico. È quindi indispensabile introdurre regole e controlli severi per prevenire il rischio di danni a persone e cose. È prioritario che il nostro paese si doti di tutti gli strumenti necessari per evitare che in futuro si verifichino tragedie 14a, Commissione ha ricordato la recente comunicazione della Commissione europea del gennaio 2009, in base alla quale potranno essere considerati compatibili con il mercato con il mercato comune gli aiuti di Stato inferiori ai 500.000 euro nel triennio 2008-2010 per le imprese che al primo luglio 2008 non si trovavano in difficoltà, estendendo questo regime anche agli aiuti

La consapevolezza dell'elevato rischio sismico suggerirebbe l'adozione di una soluzione di carattere permanente e strutturale, individuata nell'obbligo di stipulare un'assicurazione per i danni agli immobili derivanti da calamità naturale, analoga alle assicurazioni per le responsabilità civili per gli incidenti automobilistici e il rischio di insolvenza sui mutui immobiliari. Ciò permetterebbe una più equa ripartizione degli oneri per gli interventi di ricostruzione, che graverebbero in misura molto più attenuata sui singoli contribuenti. si tratta di un provvedimento importante, tempestivo e che, soprattutto, è stato concepito con l'obiettivo di non gravare ancora una volta su cittadini e contribuenti.

a noi senatori e al Gruppo del Partito Democratico di dedicare la maggior parte del tempo a disposizione per l'illustrazione degli emendamenti, nella speranza che la maggioranza possa coglierne gli aspetti positivi.

della legge di conversione del decreto-legge. È evidente che la pressione del Gruppo del Partito Democratico e degli altri colleghi dell'opposizione, insieme alle evidenti emergenze segnalate sul territorio, ha fatto sì che il Governo addivenisse a più miti consigli, in particolar modo sulle questioni della concessione dell'intero contributo a fondo perduto per la ristrutturazione della prima casa. Abbiamo fatto sì che fosse reso alternativo questo contributo al credito d'imposta, che ricordo essere stato l'unico strumento inizialmente proposto dal Governo, e al finanziamento agevolato. Oggi i cittadini possono scegliere quali di queste tre modalità utilizzare per ristrutturare la prima casa. Aggiungo che grazie ad un intervento del relatore, modulato in Aula sulla base dei nostri emendamenti, è stata inserita la norma sulla riattazione degli immobili e la zona franca urbana, rispetto alla quale è stato acquisito il principio

Le forze dell'ordine stanno facendo del loro meglio su molti fronti. Ci chiediamo se questo livello di qualità - ma ne siamo assolutamente certi - verrà garantito anche nei prossimi mesi. Non abbiamo dubbi,

a sostenere che i soldi non c'erano e che non si sapeva come trovare i fondi per riuscire a risolvere i problemi derivanti dalle conseguenze del sisma. Ci chiediamo, per fare un elenco veloce delle cose che a nostro avviso potrebbero essere oggetto di miglioramento in una collaborazione reciproca tra maggioranza ed opposizione, perché i senatori abruzzesi

i contributi per le seconde case dei residenti o per le case dei non residenti. L'Aquila e i Comuni del cratere hanno una vocazione turistica altissima; insieme ai beni culturali - che rappresenta il terzo punto - realizzano il volano dell'economia reale di quel territorio. Se dunque non si agirà su quella realtà, l'economia non ripartirà. dai beni culturali. Signor Presidente, all'Aquila e dintorni vi sono 800 immobili pubblici ed ecclesiastici e 350 privati. Tutti gli emendamenti su questi temi sono stati bocciati dalla maggioranza in 13a Commissione; non c'è verso di vedere inserito in questo provvedimento un sistema migliorativo per

del Consiglio o del commissario delegato è un provvedimento amministrativo non avente forza di legge, che vale *sic et simpliciter* fino a quando dura quell'ordinanza, che è immediatamente revocabile, modificabile anche parzialmente e non crea diritti soggettivi per i cittadini abruzzesi e per chiunque ne abbia titolo. Un atto avente forza di legge, invece, lo è; altrimenti non sarebbe stato necessario inserire al comma 2 dell'articolo 1, non solo il decreto n.

soldi alle aziende pubbliche che agiscono su servizi pubblici essenziali, come gas, rifiuti ed acqua. Oggi sono società di diritto privato, società per azioni a capitale pubblico, che non ricevono più la tariffa o la bolletta pagata.

Signor Presidente, è stata inaugurata una sola scuola sotto una tenda: nient'altro! Non si capisce il motivo per cui i sindaci dei Comuni dove insistono le scuole elementari o la Provincia non possano agire immediatamente per le riattazioni e la riapertura, previo adeguamento sismico,

la zona franca urbana. È vero, abbiamo stabilito il principio, voi lo sapete, con uno strano fastidio da parte di qualche senatore della maggioranza in Commissione, ma non ci sono i soldi. soldi. Ci sono 45 milioni sul 2009, ma voi mi insegnate che il CIPE fa entrare in vigore la norma dal 1° gennaio 2010 e quindi i 45 milioni non sarebbero utilizzati; ecco perché c'è una norma, che chiediamo venga approvata dall'Aula, che mette i soldi anche sul 2010 e sul 2011. L'ultimo punto concerne la sanità.

Però sta succedendo che il personale sanitario, dipendente dalla Regione e dalla ASL, oggi viene trasferito temporaneamente a coprire gli organici di ospedali presenti nelle altre Province, svuotando la realtà ospedaliera dell'Aquila e dei Comuni del comprensorio dell'Aquila e nessuno sa, signor Presidente, conoscendo le realtà amministrative, come e quando ritorneranno in quei posti.

all'inizio di questo mio intervento lasciatemi innanzitutto rivolgere un plauso al Presidente del Consiglio, al Governo, alla macchina della Protezione civile e a tutto il Paese che, nelle ore immediatamente successive a quelle del sisma, si è mobilitato per prestare il proprio aiuto fisico, morale ed economico ai cittadini abruzzesi, che in pochi minuti hanno visto crollare, oltre alle loro case, tutte le loro certezze. Da tutte le parti d'Italia Protezione civile, forze dell'ordine, Vigili del fuoco, misericordie, pubbliche assistenze e l'eccezionale mondo del volontariato si sono attivati da subito per soccorrere le popolazioni di quei Comuni gravemente colpiti dalle scosse sismiche, alcuni dei quali sono stati quasi totalmente cancellati; poi la macchina organizzativa si è preoccupata di far giungere sul posto generi di prima necessità, di allestire i campi di emergenza per ospitare gli sfollati, ma soprattutto di fornire sicurezza, calore umano ed il necessario supporto psicologico. Il Presidente del Consiglio, cosa mai accaduta in passato in situazioni analoghe, si è subito recato di buon mattino nei luoghi del disastro, a piè di sofferenza, per trasmettere agli abruzzesi la presenza attiva e forte dello Stato e delle istituzioni. In contemporanea, una gara di solidarietà partiva dal cuore del Paese, dal cuore di quella gente che, partecipando alle numerose raccolte di fondi ed iniziative coordinate dalla nostra Protezione civile, cercava di essere vicina e di dare il proprio sostegno a quanti, riversati nelle strade abruzzesi, avevano bisogno di ritrovare la speranza, la speranza di andare avanti nonostante tutto. Sono passati più di 40 giorni dalla scossa fatale che in Abruzzo ha provocato circa 300 vittime, migliaia di sfollati, come ricordava il senatore D'Alì, e tanta disperazione; oggi, a differenza del passato, il Governo sta continuando tempestivamente a mettere in campo tutte le iniziative volte da un lato a ridare quella speranza agli abruzzesi e dall'altro a garantire certezze per il loro futuro, per superare la fase della prima emergenza ed occuparsi dell'altrettanto delicata fase dell'emergenza ordinaria e di quella della ricostruzione. E già si dice, colleghi, che nel giro di qualche mese molte persone potranno lasciare lo stato precario delle tendopoli e trasferirsi in villaggi organizzati per cercare di iniziare a riprendere in condizioni di quasi normalità la loro vita. In questo senso va il presente decreto-legge, in questo senso va la scelta fatta dal presidente Berlusconi e la tempestività delle sue iniziative, così come in questo senso va un'altra iniziativa avallata da tutti i potenti del mondo, da tutti quelli che hanno avuto la forza di avallare un'iniziativa del presidente Berlusconi, che ha molto colpito l'opinione pubblica e tutti noi: quella di trasferire il G8 dalla sede della Maddalena alla città dell'Aquila. È un sacrificio che può certamente apparire di poco conto se paragonato agli indubbi vantaggi che possono trarne le popolazioni abruzzesi che oggi vivono in difficoltà infinitamente maggiori di quelle dei miei conterranei; un sacrificio che sono convinto che, al di là della delusione e dell'amarezza dei maddalenini, dei galluresi, dei sardi, al di là delle delle preoccupazioni sullo stato e sui tempi delle opere in corso di realizzazione e su quelle da realizzare, al di là del lungo elenco delle occasioni sfumate, rappresenta il pegno della solidarietà e della necessità che occorra contribuire immediatamente al rilancio socioeconomico dei territori colpiti dal sisma. È un sacrificio che, sono convinto, i sardi porteranno avanti con onore, con quella grandezza d'animo e generosità che ci contraddistingue. Ma per capire la legittima delusione e le preoccupazioni dei sardi, colleghi, bisogna scavare indietro nel tempo, in quei cento e più anni di servitù militari che hanno pesantemente condizionato lo sviluppo dell'isola della Maddalena e in questi ultimi vent'anni passati a dibattere su possibili su possibili modalità di una riconversione, in questi ultimi anni trascorsi rincorrendo la speranza che il G8 potesse rappresentare quella occasione a lungo inseguita per il rilancio, lo sviluppo e la valorizzazione dell'isola. Colleghi, anche in questa terra ci è voluta la presenza dello Stato, l'azione incisiva del Presidente del Consiglio e l'efficienza della macchina organizzativa della nostra Protezione civile, tra le migliori al mondo, che hanno saputo, in soli nove mesi, che hanno saputo, in soli nove mesi, cambiare il volto ad un territorio, effettuando grandi opere di risanamento ambientale e trasformando quei luoghi pesantemente danneggiati dalla presenza militare in un polo di eccellenza turistica. Colleghi, ieri ho effettuato un sopralluogo nei cantieri, ormai quasi totalmente avviati a conclusione. Essi rappresentano un esempio di eccellenza, un vanto per la Sardegna e per il Paese intero. I sardi oggi oggi chiedono soltanto una cosa: che non vengano dimenticati, che tutti gli impegni assunti dal Governo vengano mantenuti. colleghi, consentitemi di rivolgere un plauso ai cittadini abruzzesi per la dignità e la forza d'animo con cui hanno affrontato e stanno affrontando la situazione di emergenza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, lo scorso 6 aprile il terremoto ha devastato la bellissima terra d'Abruzzo e cambiato indelebilmente la vita dei suoi cittadini. Da questa tristissima esperienza è emersa la parte migliore dell'Italia, la fierezza e la dignità del popolo abruzzese, la tempestività degli aiuti dei vigili del fuoco, delle tante associazioni di volontariato e della Protezione civile, la solidarietà di cittadini comuni che hanno voluto, secondo le proprie possibilità, aiutare le persone colpite. Oggi desidero pubblicamente ringraziare di cuore quanti hanno collaborato e che ancora si impegnano ogni giorno sullo straziato territorio abruzzese. Anche se è passato già del tempo, voglio ricordare le 299 persone che hanno perso la vita in quella terribile notte e ricordare soprattutto i numerosi giovani che sono morti nella Casa dello studente per l'incuria e la superficialità di chi avrebbe dovuto effettuare i controlli e tener conto di quanto già avevano denunciato i ragazzi prima di quella notte e non l'ha fatto. Voglio ricordare quella gente che è morta perché in una zona sismica la logica del guadagno, purtroppo, ha prevalso sulla necessità di attenersi a norme ben precise. Ora, anche in memoria di chi ha perso la vita, passata la fase dell'emergenza, bisogna fare in modo che i cittadini dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal sisma ritornino a vivere e recuperino la loro quotidianità. È necessario che si cominci a pensare alla fase successiva alle tendopoli, che si faccia in modo che le imprese riprendano la loro attività, che a settembre ci siano vere scuole e strutture universitarie ad attendere i ragazzi. Il provvedimento in esame, sebbene migliorato lievemente in Commissione, continua a dimostrarsi insufficiente. Le tendopoli si stanno dimostrando inadatte anche dal punto di vista igienico-sanitario già al primo innalzamento delle temperature. Possiamo immaginare cosa diventerà nel pieno della stagione estiva e, ancora peggio, quando in inverno arriveranno il freddo e la neve. I più a rischio sono gli anziani e i malati costretti a letto, per i quali è necessario provvedere subito con sistemazioni più idonee. Bisogna agire in fretta, fare in modo che le case lesionate vengano rese agibili, che si cominci a pensare alla ricostruzione di quanto è andato distrutto - non certo alla costruzione di un'altra città stile Milano 2, che qualcuno ha menzionato - e che si pensi a sistemazioni valide nella fase di passaggio. Per fare questo, è necessario che ci siano soldi veri e in tempi brevi. Siamo soddisfatti che in Commissione sia passato il principio che i cittadini abruzzesi valgono quanto quelli di Umbria, Marche o Friuli, vittime della stessa terribile esperienza, e che quindi gli indennizzi del danno subito siano del 100 Ma i fondi stanziati non sono sufficienti e soprattutto nulla è stato previsto per l'immediato, per il 2009. È prioritario, dicevo, e anche altri colleghi lo hanno sostenuto, aiutare le imprese a riavviare le attività imprenditoriali e commerciali, per fare in modo che gli aquilani tornino a lavorare, facilitando il riavvio delle imprese, anche utilizzando prevalentemente quanto prodotto dalle popolazioni locali. Immagino abbiate visto in televisione i litri di latte buttati dagli agricoltori locali o la carne tedesca utilizzata per le mense delle tendopoli. Tra l'altro, dopo i tanti annunci, resta il problema che il Governo assicura la copertura di indennizzi ai lavoratori precari e autonomi rimasti senza lavoro solo per tre mesi e per quelli che hanno diritto alla cassa integrazione una proroga di solo sei mesi. Anche le notizie sulla scuola non sono certo confortanti: i tagli di organico previsti dal decreto Gelmini non risparmieranno l'Abruzzo, per il quale non è prevista alcuna deroga, e parte dei soldi da investire per le scuole abruzzesi sono gli stessi, cioè pochi, previsti per gli interventi in tutta Italia. Ricordiamoci, inoltre, che una voce importante dell'economia aquilana risiede nella sua vocazione universitaria, visto il grande afflusso di studenti dalle vicine Regioni centro-meridionali e anche dall'estero. Per questo è necessario prevedere, prima della ripresa dell'anno accademico, una sede alternativa per la casa dello studente e per l'università, utilizzando anche le caserme rimaste illese. Come consigliato da una delegazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha portato il contributo della propria esperienza in Abruzzo, è necessario che la ricostruzione venga fatta rapidamente, con la massima trasparenza sui fondi erogati, con un controllo amministrativo centrale e la partecipazione attiva della popolazione, coinvolgendo in tutte le fasi i sindaci dei Comuni interessati e i Presidenti della Provincia e della Regione. Ieri ero all'Aquila e dai cittadini ho raccolto delle specifiche richieste, di cui sono oggi portavoce. Le piccole imprese commerciali chiedono che sia previsto dal Commissario delegato che gestisce i fondi un indennizzo per le merci deteriorate e un contributo per l'acquisto di nuovi frigoriferi per lo stoccaggio delle scorte. Inoltre, si sollecita un piano che preveda, per la riapertura degli esercizi commerciali, affitti a canone agevolato e crediti garantiti. Richieste sono arrivate dai comuni cittadini che sollecitano un sostegno psicologico continuativo da parte di esperti. Inoltre, le famiglie residenti negli alberghi sulla costa, anche per rispondere alle richieste degli albergatori che vorrebbero riprendere l'attività turistica, chiedono la possibilità di un contributo diretto per provvedere autonomamente ad una sistemazione, cosa che tra l'altro risulterebbe più economica. Non condividono, invece, la proposta di spostare il G8 all'Aquila: è un gigantesco spot pubblicitario, che non aiuta la popolazione, ma ingigantisce i problemi intralciando i lavori di ricostruzione. Sono certa che il testo arrivato in Aula, con la collaborazione e la disponibilità di tutti, si possa ancora migliorare. L'Abruzzo è scomparso dalle notizie sui quotidiani, ma facciamo in modo che non cali la nostra attenzione e non manchino risposte chiare ed efficaci ai problemi degli abruzzesi.

e chiedo scusa a lei e ai colleghi se non riesco ancora a convertirmi alla dottrina del «tirare a campare» o del «chi te lo fa fa'». Forse è un segno di giovinezza residua.

di quanto il sottoscritto e numerosi altri senatori hanno inteso fare, dire e ottenere. Sarò un po' più preciso.

aventi ad oggetto la competenza che il testo base intendeva spostare sulla procura della Repubblica del capoluogo di distretto

sul quale, oltre che sugli emendamenti a mia firma, mi sono permesso di riprendere la parola, richiamando sommariamente gli argomenti che avevo già svolto e segnalando alla Presidenza che non era proceduralmente

Dirò di più: di fronte a qualche incertezza da parte del Governo e del relatore in ordine a tale argomento di natura specifica, che non travolgeva certamente l'impianto della legge che stavamo discutendo ma che era di notevole importanza, prese la parola anche un collega dell'opposizione, precisamente il senatore Casson, corroborando i miei argomenti e chiedendo una votazione per parti separate, perché effettivamente un conto era l'insieme dell'articolo ‑ come si andava ad emendare ‑ e altro conto erano le proposte che si andavano ad incentrare

ma successivamente il Presidente pose ai voti, secondo ciò che io e numerosi altri senatori intendemmo, la soppressione dei commi 4 e 5, giusta dunque i miei emendamenti 9.304 e 9.305. invece, rilevo che si intese mettere ai voti il testo quale era nell'emendamento del relatore, e dunque praticamente il testo base.

praticamente quasi tutti o comunque numerosi senatori, tant'è che essendo stati votati praticamente all'unanimità (noi tutti compresi, compreso il presentatore degli emendamenti soppressivi, cioè il sottoscritto) per alzata di mano, si disse che erano approvati. Autorevoli senatori della maggioranza e della minoranza, come sempre avviene scherzosamente nel costume parlamentare, si congratularono con me e dissero: «Stasera dovrai pagare un ricco aperitivo». Per la verità, a me personalmente non me ne veniva niente: rimediavo solo ad un madornale errore con cui abbiamo ingolfato ulteriormente le procure distrettuali della Repubblica, creando un pasticcio di cui evidentemente poco interessa a chicchessia.

che dico - che alla Camera è andata un'altra faccenda, e precisamente è stato ribadito il testo base con il maxiemendamento del relatore, come se non avessimo fatto nulla. Da ciò derivano le mie rimostranze e l'espressione della mia amarezza.

Allora, se c'è il verbale posso togliermi i sonagli dal berretto. La risposta burocratica non accontenta me e i senatori che intendevano, su parere unanime della Commissione giustizia, legiferare diversamente. Non oso sperare che i colleghi della Camera rettifichino questo grave errore e questo grave inconveniente procedurale. Non oso sperarlo, non sono più nell'età delle speranze. Voglio però sottolineare e lasciare a verbale tutto questo per ogni seguito. E desidererei che, anche nei momenti congestionati delle sedute, la Presidenza si regolasse in maniera tale

attingerlo. In qualche modo intendo, sia pure con il massimo rispetto verso la Presidenza, lamentarmi sentitamente dell'esito legislativo di questa complessa procedura e sperare che vi siano margini e circostanze per potervi rimediare.

e poi la restante parte dell'emendamento, di cui facevano parte quei due commi. L'Assemblea, visto il parere cui lei faceva riferimento, avrebbe dovuto in quel momento respingere questi due commi; è chiaro che

Presidente, rispetto profondamente le convinzioni del collega Benedetti Valentini, perché so con quanta passione è intervenuto più volte su tali aspetti,